Comunico che, in data 14 agosto 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle rispettive deleghe di funzioni conferite dai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso i medesimi Dicasteri sen. Vito Claudio CRIMI, on. dott. Matteo MAURI,

«Onorevole Presidente, informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca il dott. Giuseppe DE CRISTOFARO, con la cessazione contestuale dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Istruzione. Con viva cordialità, *f.to*Giuseppe CONTE». In data 14 agosto 2020, sono stati presentati i seguenti disegni di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:* «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020» *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»

più costruttivi e più cospicui. Vorrei portare all'attenzione di tutti, soprattutto del Presidente della Regione Lazio e del ministro Speranza, l'idea del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, e dei consiglieri comunali di Fiumicino D'Intino e Poggio, di realizzare una struttura sul litorale di Roma Nord che comprenda tutti i Comuni limitrofi; si tratta di

da terrorismo psicologico e psichico nei confronti delle persone, con questo Covid che sembra oramai perdurare e non finire mai (l'altro giorno abbiamo letto di questa ordinanza), riteniamo che le strutture sanitarie debbano essere serie e non delle prese in giro per i cittadini. Fiumicino, Ladispoli e Cerveteri meritano un vero ospedale, non delle banali bufale

Signor Presidente, intervengo per fare uno dei lavori che gli italiani non vogliono più fare, in particolare gli italiani di maggioranza, cioè richiamare il Governo al rispetto degli impegni presi con il Parlamento. Ricordo che la risoluzione n. 1 (testo 2), approvata nella seduta del 28 luglio 2020, dopo aver premesso che non vi erano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali e aver richiamato l'esigenza di rispettare la proporzionalità nelle misure di contrasto all'epidemia, invitava il Governo a definire con norma primaria le eventuali misure di limitazione delle libertà fondamentali e assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative dello stato di emergenza. Questo non era semplicemente un impegno che il Governo prendeva con il Parlamento, ma era anche il preciso disposto dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che imponeva al Presidente del Consiglio dei ministri (o a un Ministro da lui delegato) di riferire preventivamente il contenuto dei

Consiglio dei ministri che poi deve intervenire, come del resto la stessa ordinanza del ministro Speranza precisa. Le condizioni di particolare urgenza rendono ancora più cogente l'obbligo di motivare e documentare la proporzionalità. Noi abbiamo 2020 - che, nonostante incida su libertà fondamentali come quella di circolazione, non solo non è per definizione una norma primaria ma addirittura, seguendo un malcostume dell'attuale Governo, interviene sovvertendo la gerarchia delle fonti impone una deroga a quanto stabilito nella norma primaria, ovvero il fatto che le Regioni possano intervenire sui provvedimenti del Governo in senso sia ampliativo che restrittivo. Invece, per Speranza si può solo essere più severi di Speranza.

per valutare la proporzionalità di questo intervento così rigoroso. Quindi, più in generale, non viene spiegato il motivo dell'estrema necessità e urgenza. Devo dire che del parere del CTS (che, ricordiamocelo, ci aveva promesso 151.000 ricoverati in terapia intensiva il 28 aprile 2020)

che il signor Ministro venisse a riferire, come richiesto dal decreto-legge n. 19. *(Applausi)*, e in particolare che ci desse dei dati per valutare la proporzionalità dell'intervento cosa che questa maggioranza ha chiesto di poter fare.

Se li ha, il Ministro deve darli perché ha preso l'impegno di farlo con il Parlamento; se non li ha, sarebbe meglio che si astenesse, per il futuro, da questi spregiudicati interventi normativi.

e irriverenti posti in essere da un rappresentante dell'opposizione del quale non farò il nome (ma certamente chi mi ascolta capirà a chi mi sto riferendo). Signor Presidente, il negazionismo è il peggior male di questi tempi. Il *trend* in aumento dei contagi da Covid ci spinge a sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare i giovani, al rispetto rigoroso della normativa sul distanziamento sociale, o almeno questo è quello che la logica invece, c'è chi, in perenne campagna elettorale e nell'attesa dei pieni poteri, non solo esprime e propaganda il negazionismo, ma lo pratica anche. È dal 2 giugno scorso che siamo costretti a subire assembramenti, in totale spregio delle norme sul distanziamento sociale, per un singolare capriccio dovuto alla necessità di tornare in campagna elettorale (fatta di *selfie*, anche questi irriducibili e irriverenti). Tutti i cittadini sono stati e continuano a essere molto attenti affinché il virus non torni a prevaricare sulle proprie vite. Il *lockdown* è servito proprio a questo, ma a un certo punto qualcuno ha deciso di essersi stufato di questo distanziamento sociale ed è tornato a creare assembramenti per strada e a mettere se stesso e gli altri a rischio di contagio. Usare una falsa politica, quella negazionista, che di politico ha davvero ben poco ed è una totale prevaricazione sugli altri, solo questo, è avvertito come una minaccia per tutti. I cittadini che credono ancora nelle istituzioni ci chiedono a gran voce che tutti siano soggetti alla medesima legge. Non è possibile che un comune cittadino se non rispetta il distanziamento sociale è soggetto a multe mentre se lo fa un rappresentante della politica ne ne risulta esentato. Chiedo attenzione su questo tema, signor Presidente, perché non è un mio capriccio, ma si tratta di sfatare quel senso di diseguaglianza nell'applicazione della legge, diseguaglianza percepita dal cittadino, che è stato rigoroso e che continua a esserlo, ancora oggi, collaborando con lo Stato. La legge è uguale per tutti. Questo è un dogma, è un principio fondamentale. Perché, allora, le sanzioni le subiscono solamente i cittadini comuni e non quei politici che amano

le regole e «se lo fa lui, posso farlo anche io»; è questo quello che dicono ed è questo quello che poi fanno. Siamo a ridosso della riapertura delle scuole e stiamo vivendo una fase particolare in cui le attività ricettive danno il loro meglio per evitare il peggio. Stiamo facendo tutti dei grandi sforzi e qualcuno ha l'irriverente coraggio di annullarli completamente. Signor Presidente, noi abbiamo due nemici invisibili oggi: uno si chiama Covid-19 e l'altro si chiama ignoranza.

Senatore Bagnai, le faccio presente che lei ha usato aggettivi ben più problematici. La prego di accomodarsi

Signor Presidente, dopo aver abolito il Comitato per le questioni degli italiani all'estero e avere impedito agli italiani all'estero di eleggere a fine scadenza le proprie rappresentanze Comites, dopo averli dopo averli obbligati a pagare l'IMU sulle case che hanno in Italia come se fossero seconde case, dopo aver loro imposto di votare all'estero, dove ci sono più di 20 consolati che non sono in grado di offrire

di violazione dei diritti degli italiani all'estero. Si tratta di una diminuzione della rappresentanza che abbiamo più volte denunciato in questa sede, con quattro senatori in rappresentanza di sei milioni di italiani all'estero. Noi abbiamo, *ictu oculi*, segnalato che non c'è una democrazia nel mondo che abbia come rappresentanti quattro senatori eletti in un collegio di sei milioni di persone.

è stato rigettato qualche giorno fa per mancanza di legittimità, non in quanto io senatore avvocato ma in quanto non avrei subito gli effetti pregiudizievoli di questa riforma. È un po' come dire a qualcuno che segnala che c'è un pazzo che passa con il rosso

con legge costituzionale si deciderà di porre in schiavitù gli italiani all'estero (faccio una provocazione, ma il ragionamento purtroppo fila), cioè quando una legge costituzionale palesemente incostituzionale, a scapito di cittadini di serie B come siamo noi italiani all'estero, verrà approvata dal Parlamento e qualcuno si rivolgerà in ultima analisi alla Corte costituzionale e gli verrà detto che non è legittimato, in quanto ancora non è stato fatto schiavo, in quel momento le garanzie per i cittadini italiani all'estero saranno finalmente riconosciute *(Applausi)* o si continuerà ad andare avanti su questa strada ignobile, in cui noi siamo trattati come cittadini non di serie B, ma di serie C o di serie D, D, senza che le prerogative costituzionali di questo Parlamento e di altri organi di rilievo costituzionale, *in primis* la Corte costituzionale, possano avere effetto? Questa è una denuncia io mi appello, in ultima analisi, a tutte le più alte cariche dello Stato per cercare di bloccare *in extremis* questa gravissima violazione dei nostri diritti politici.

previsto dal Governo per aiutare i detentori di partite IVA che stanno vivendo una difficoltà economica determinata dal coronavirus. Il MoVimento 5 Stelle ha condannato questi atteggiamenti e ho accolto con favore l'invito del capo politico Vito Crimi di

mi ha fatto molto piacere sentire in questi giorni e apprendere dalle notizie di stampa che il senatore Salvini, segretario della Lega, ha tuonato contro questi furbetti, affermando che avrebbe utilizzato il pugno duro, a partire dal divieto di ricandidabilità dei rappresentanti della Lega che abbiano chiesto e ottenuto questo *bonus* senza averne diritto.

non di prendere per certo e per vero quello che sto dicendo, che apprendo dagli organi di stampa, ma di appurare egli stesso, chiamando ad esempio il sindaco leghista del Comune di Potenza e chiedendogli informazioni, spiegazioni e chiarimenti riguardo a due assessori della Giunta leghista del Comune di Potenza,

che deriva dalle *royalties*. Viggiano è un Comune sul quale insistono pozzi petroliferi e il tristemente noto COVA di Viggiano, che è un centro oli. Stando poi agli articoli di giornale che sono usciti stamattina (di cui riporto velocemente uno stralcio), pare che abbiano usufruito di questo *bonus* lo stesso sindaco, i fratelli, alcuni familiari e il cognato; pare che abbiano usufruito di questo *bonus* anche membri della Giunta (un suo assessore e il suo capogruppo) e pare che abbia firmato questa delibera lo zio del sindaco. Secondo le spiegazioni e le giustificazioni che ha dato il sindaco, pare che sia tutto legittimo e io voglio crederci. Ma vorrei dire al senatore Salvini, che appurerà sicuramente quanto riportato, che esiste anche un diritto non scritto, una legge che si rifà semplicemente all'etica